Vengono quindi semplificati molti adempimenti burocratici per l'accesso ai fondi antiracket e antiusura. Indubbiamente anche questo rappresenta un passaggio estremamente importante del provvedimento.

che offre alle famiglie, ai singoli consumatori ed anche alle piccole imprese, oggi escluse dall'assoggettabilità alle procedure fallimentari, la possibilità di trovare uno strumento trasparente ed efficace per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento e delle crisi di liquidità dovute a situazioni di squilibrio economico fra le obbligazioni e gli impegni precedentemente assunti e il reddito ed il patrimonio disponibili. Ho già indicato ieri molte legislazioni europee che contengono uno strumento di questo tipo. L'Italia, purtroppo, fino ad oggi non si è mai dotata di una procedura trasparente

in particolar modo alla mancanza degli incentivi fiscali volti a rendere ancora più importante e allettante anche la procedura per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento. Crediamo

che immaginiamo trovi il consenso di tutte le parti politiche. Ora sta al Governo utilizzare questo importante strumento, anche anticrisi, magari dotandolo di quegli incentivi fiscali necessari per farlo decollare.

e per aver evidenziato l'importanza di questo provvedimento dal punto di vista sistematico, inquadrandolo in un'ottica di sistema, provvedimento che consente di svolgere un'azione più efficace nella lotta a questi due gravi fenomeni dell'estorsione e dell'usura. Non posso che ringraziare ancora dei contributi offerti. Ritengo che questo disegno di legge, ribadisco, di iniziativa parlamentare, potrà dare una soluzione efficace ad un problema sentito particolarmente in un momento di grave crisi economica.

che questo provvedimento, licenziato dalla Commissione con un accordo quasi unanime e con un contributo dell'opposizione, evidenzia una

Bisogna dare atto al presentatore, senatore Centaro, di aver portato la questione all'interno del Parlamento, per un'iniziativa parlamentare, forse la prima che in questa legislatura trova un consenso unanime.

Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.200 e 3.0.200, sulle quali il parere è contrario,

che è bene che venga affrontata all'inizio dell'esame di un disegno di legge il cui Capo II è interamente dedicato al sovraindebitamento delle famiglie in chiave di prevenzione antiusura. Da tempo le associazioni chiedono una riforma della legge n. 108 del 1996 che assicuri anche alle famiglie, come accade per gli imprenditori, l'accesso al Fondo di solidarietà. Questo emendamento va proprio in tale direzione.

integrando la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. La Commissione giustizia, nell'apportare modifiche al testo originario del disegno di legge, ha inteso affermare il criterio della particolare attenzione per i requisiti soggettivi dei destinatari dei mutui, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della 1.203, anch'esso approvato dalla Commissione giustizia, stabilisce con rigore che l'erogazione dei mutui all'imprenditore individuale dichiarato fallito trova un ostacolo non solo nella condanna per reati fallimentari o contro il patrimonio, ma anche nella circostanza che egli risulti imputato o persino solo indagato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui è sospesa fino all'esito dei all'emendamento 1.208, il testo approvato dalla Commissione prevede che le riunioni della commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura «sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate». Il testo prosegue stabilendo che «le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti». Ebbene, appare opportuno non confondere il *quorum* per la validità della riunione con quello deliberativo

in effetti si tratta di un emendamento che ripete la stessa dizione approvata dalla Commissione,

in Commissione giustizia. Si tratta di una cautela che trova fondamento nell'opportunità di assicurare che i fondi a disposizione che ovviamente non saranno infiniti - non vadano a soggetti la cui condotta imprenditoriale abbia integrato ipotesi di reato strettamente connesse all'attività di impresa. Il testo, così com'è oggi, limita però i casi alla bancarotta: con questo emendamento si intendono invece prendere in considerazione tutte le fattispecie di cui al Titolo VI della legge fallimentare,

coerenza del sistema delle pene previste dal nostro codice;

pesantissimi in termini di libertà e di vite umane, che l'organizzazione mafiosa è una minaccia particolare che tocca la radice della nostra convivenza sociale, economica e economica e democratica. Ecco perché nel 1982 - lo ricordo ai colleghi ‑ quando fu inserito il reato di associazione mafiosa,

della tradizione del nostro ordinamento democratico, della migliore cultura giuridica del nostro Paese. Eppure, allora si fece una scelta intelligente, certo limitata perché

questo particolare provvedimento, cadde il 3 settembre. Il Parlamento arrivò dopo e fu quella una grande innovazione che inserì in sostanza un'idea moderna, un sistema di cosiddetto doppio binario, che poi via via si articolò sia sul piano delle norme penali sostanziali sia procedurali, sia anche nell'organizzazione del nostro ordinamento. Faccio un esempio: pensate alla DDA. Quando Falcone pensò a questo sistema ci furono legittime e motivate idee di resistenza e di opposizione, nonché conflitti all'interno dello stesso mondo della magistratura; eppure fu una grande intuizione di cui oggi, grazie all'idea di Falcone, raccogliamo ottimi risultati.

Il più delle volte con gli stessi affiliati che fanno capo alla stessa famiglia; c'è un *turnover* impressionante nell'organizzazione delle attività criminali che attengono sempre alle stesse persone, al massimo alla stessa famiglia, che nel giro di quattro‑cinque anni riescono ad uscire fuori dal carcere, riprendono immediatamente l'iniziativa e lo Stato deve prontamente provvedere alla riorganizzazione di una delle più costose e pericolose attività di indagine e processuali per ottenere poi lo stesso risultato, ovvero colpire la stessa persona, al massimo la stessa famiglia. Allora, c'è da fare una riflessione se questi sono i risultati: è possibile inserire un sistema di doppio binario che, al pari di altri ordinamenti,

Penso che una riflessione vada avviata e per questo ho presentato questi emendamenti, che mi auguro l'Assemblea cominci a valutare non secondo lo schema della coerenza con il nostro sistema giuridico e penale; infatti, anche allora quando si opposero queste motivazioni non si capì la specificità e la minaccia particolare che l'organizzazione mafiosa porta alla nostra convivenza, alla democrazia e al nostro sistema delle libertà.

ed ha una forza in sé), riprende il suo cammino e torna a mettere in ginocchio, soprattutto con il sistema dell'estorsione e dell'usura, il nostro sistema economico e produttivo. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti del Centro di formazione professionale ENAIP Trentino di Trento. A loro rivolgiamo un saluto e gli auguri per la loro attività.

Nel caso in specie, all'articolo 629 è stata introdotta una specifica aggravante qualora il fatto estorsivo sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari. È evidente che questo è già una presa di posizione positiva, che manifesta la volontà di punire maggiormente le condotte delittuose legate all'usura. Però occorre prendere atto - e credo anche coscienza del livello ormai professionale che le dinamiche estorsive hanno assunto, anche in riferimento alle organizzazioni criminali mafiose e soprattutto del giro di affari connesso a questo fenomeno, particolarmente capillare in talune aree del nostro Paese. Paese. Con l'emendamento 4.201 si propone di alzare significativamente il livello della sanzione. Il carattere organizzato della dinamica estorsiva che porta all'accumulo di ingentissime quantità di denaro destinate al riciclaggio emerge anche nelle aree di più recente insediamento mafioso, ovvero in quelle dove il criminale non ha l'assoluta certezza della rassegnata omertà delle vittime, e consiste in una inversione della relazione richiesta-intimidazione. Dal punto di vista della mafia l'estorsione si trasforma quindi in un vero e proprio servizio di protezione sollecitato dalla vittima. Il secondo elemento di novità che possiamo rilevare nell'organizzazione del fenomeno e che ci porta a richiedere questo inasprimento della sanzione è è quello della orizzontalizzazione della pratica estorsiva. L'organizzazione mafiosa punta ad una estensione del numero dei soggetti da contattare imponendo dazioni di modesta entità: pagare poco, ma pagare tutti. L'esito complessivo delle entrate resta assolutamente ingente, ma si raggiunge l'ulteriore obiettivo di ramificare un controllo più pregnante delle aziende, un controllo più pervasivo soprattutto delle piccole e medie aziende. Possiamo quindi dire che la mafia si è venuta configurando come un sistema criminale apparentemente compatibile con il settore economico aggredito. Aggiornare le sanzioni al livello del sistema finanziario estorsivo, intimamente connesso all'usura, credo sia dunque una scelta condivisa volta a rafforzare l'intero apparato sanzionatorio anche sul fronte delle aggravanti.

Abbiamo inteso farlo attraverso una estensione degli strumenti della protezione processuale della parte offesa, previsti in linea generale nel nostro ordinamento, anche alle fattispecie dell'usura e della estorsione. È del tutto pacifico che l'effetto mediato del potenziamento di questi strumenti di protezione processuale sarà quello del potenziamento del contrasto criminale in linea generale, anche a seguito di un'automatica e conseguente maggiore induzione alla denuncia da parte delle persone offese e, quindi, al contributo perché queste si liberino dello stato di sottomissione

abituali e sono maggiormente indotti a ricorrere a scorciatoie, ci è sembrata assolutamente opportuna. Per non intervenire in maniera assolutamente asincrona rispetto al sistema, abbiamo mutuato l'intervento dal sistema processuale di protezione già ordinariamente esistente che riguarda i minori di età e le persone sottoposte a violenza sessuale. Passo rapidamente in rassegna le disposizioni che nei sette commi di cui è composto il proposto nuovo articolo 5‑*bis* del disegno Il comma 1 prevede l'estensione della possibilità di ricorrere all'anticipazione dell'assunzione della prova al momento delle indagini preliminari attraverso l'incidente probatorio, estendendo anche alle fattispecie previste dagli articoli che riguardano l'usura e l'estorsione le facoltà relative alle violenze sessuali e alle violenze nei confronti dei minori.

Il comma 3 richiama l'articolo 472 del codice di procedura penale e quindi estende anche a queste fattispecie uno strumento tipico di protezione quale è quello dell'ascolto della persona offesa il sistema delle porte chiuse. È un potente strumento di assistenza psicologica nei confronti di una persona che, nel quadro della commissione del reato, ha assunto, non solo il ruolo della persona offesa, ma anche, torno a ripetere, quello della persona sottomessa dal punto di vista psicologico. Così pure il comma 4, che si riferisce all'articolo 190-*bis* per i colleghi che hanno un meno dimestichezza con il nostro codice di diritto penale posso dire che il comma estende anche a queste fattispecie il meccanismo che impedisce la reiterazione della prova già raccolta in contraddittorio, sempre inutile e a volte potenzialmente molto pericolosa.

il magistrato procedente ne ravvisa l'opportunità), attraverso il sistema del cosiddetto vetrospecchio e dell'audizione a mezzo di citofono, quindi per impedire un contatto diretto tra la persona offesa e la persona che ha recato l'offesa. I commi 6 e 7 sono un potenziamento processuale importante. processuale importante. L'articolo 406 estende anche a queste fattispecie la possibilità di prorogare i termini delle indagini per il pubblico ministero, peraltro esentandolo dal notificare all'indagato la richiesta di proroga. che riguardano i fenomeni di usura e di estorsione sono a volte molto complicati e devono trovare la loro traccia prima e il consolidamento della prova dopo, solo attraverso analisi di moltissimi documenti, soprattutto di natura bancaria, quindi a volte di difficile comprensione.

un meccanismo di richiamo determini l'aumento anche del periodo di massima custodia cautelare. Vorrei aggiungere, Presidente, se lei me lo consente, una breve riflessione sull'emendamento successivo, 5.0.201, presentato dai colleghi Casson, Carofiglio e altri,

riguarda l'estensione della possibilità di assumere l'incidente probatorio anche con riferimento alle dichiarazioni discordanti o alle dichiarazioni rese in altro incidente probatorio,

che sono quelle che in una sorta di cascata derivano dall'applicazione del comma 1-*bis* dell'articolo 392, che è richiamato dal 393, comma 2-*bis*, richiamato dall'articolo 398, comma 3-*bis*. Riguarda questa disposizione il deposito degli atti da parte del pubblico ministero, la cosiddetta *discovery*, quindi sono aspetti importanti del processo.

a cui rinnovo l'invito a riconsiderare questo aspetto.

e di una formulazione che tiene conto del pericolo di intimidazioni che si possono verificare nei confronti delle persone che dovrebbero rendere dichiarazioni possibilmente in sede dibattimentale, ma anche durante la fase delle indagini preliminari mediante lo strumento dell'incidente probatorio.

Da un punto di vista contenutistico riteniamo che questa impostazione sia processualmente quella più ampia e corretta proprio perché riguarda tutte le fattispecie di persone che dovrebbero essere sentite mediante lo strumento probatorio.

5.0.200 (testo 2), con l'aggiunta delle ulteriori possibilità di incidente probatorio nel caso del contrasto con altre dichiarazioni o con altro incidente probatorio. In questo caso sono d'accordo

per i delitti di cui agli articoli 644 o 629 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti"».

Sinceramente, non comprendo quest'ultimo intervento. C'è l'accordo del Governo, del relatore

Si tratta di disposizioni che si legano l'una all'altra in un sistema complesso; pertanto consentire al relatore di riscrivere la norma dopo aver fatto tutti i coordinamenti è un principio di precauzione che il senatore Ferrara intelligentemente suggerisce.

Il problema era di rendere possibile egualmente il patteggiamento della pena sotto il profilo della deflazione del processo penale, subordinandolo però assolutamente al risarcimento del danno: ciò tutela la vittima e, nello stesso tempo, rende più rapido il processo.

perché riguarda ancora una volta la tutela delle persone offese vittime dei reati di usura e di estorsione. Si tratta di una norma che interviene in materia di testimonianze, che in questo caso possono essere rese

8.0.201, che riprende, con riferimento all'usura, alcune considerazioni che il procuratore nazionale antimafia aveva svolto in sede di audizione sul disegno di legge n. 733, riguardante misure di sicurezza pubblica. Con il comma 1 proponiamo di intervenire sul codice dei lavori pubblici al fine di stabilire che, ovviamente fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione antimafia, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché ancora per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento possa proporre alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento,

dia comunicazione alla polizia tributaria e all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'applicazione di quanto di loro competenza, quando esercita l'azione penale per i delitti di cui all'articolo 629 (estorsione) e 644 (usura) del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378 e 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti di attività commerciali.

e tutelare meglio le persone offese dai reati di estorsione e di usura e che abbiano reso dichiarazioni o comunque fornito elementi funzionali all'individuazione dei soggetti autori dei fatti criminosi. È evidente che questo nasce dalla circostanza della difficoltà dell'accertamento della condotta illecita e del reato, e quindi dei soggetti autori. Infatti le condizioni, anche di natura ambientale, nell'ambito delle quali si sviluppa e si realizza la condotta illecita, sono tali da non mettere il soggetto passivo del reato nelle condizioni di poter sempre denunciare, soprattutto nel momento in cui si trova in una situazione di inferiorità economica di particolare natura e rilievo. Sicché, credo sarebbe opportuno consentire in questa ipotesi la possibilità di avere una serie di incentivi, anche di natura fiscale, che poi sono quelli che interessano all'operatore economico nel momento in cui cerca di evitare il doppio danno dai reati di estorsione o di usura, cioè il danno del

quindi ai cittadini che non svolgono attività imprenditoriale, e ai piccoli imprenditori che non rientrano nelle procedure concorsuali. quindi, che l'approvazione dell'emendamento 10.202 limita fortemente la platea delle persone che possono usufruire di questa procedura, imprenditoria o di attività commerciale in forma societaria operiamo un'ulteriore restrizione anche nell'ambito dell'imprenditoria.

prevede l'opportunità (e non la necessità) che nel cosiddetto piano di rientro l'azione possa essere messa in capo ad un unico soggetto mediante normale cessione del credito. Si tratta di un'opportunità

anche un'attenzione importante sulle ulteriori possibilità per la persona in difficoltà di accensione di nuovi finanziamenti e soprattutto dell'utilizzo di taluni strumenti di pagamento elettronico: ci riferiamo in particolare alle carte *revolving*, che sono uno dei motivi per cui diverse famiglie entrano in difficoltà. Pertanto, a nostro avviso è molto importante che venga posta attenzione sulla limitazione di ulteriori finanziamenti e accessi al credito nel piano di rientro. PRESIDENTE.

al parere del Governo.

Il parere del Governo

nascono da un'esigenza relativa all'impostazione dell'articolo 18 che tratta di organismi di composizione della crisi e, in e, in particolare, degli enti che dovrebbero essere abilitati a costituire tali organismi dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità

con situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e con questioni di usura. Pertanto, proprio per la serietà dell'istituto, riteniamo che la dizione «enti pubblici» vada limitata, oltre ai casi già indicati dal comma 4,

Ogni collega è pregato di votare per sé. **Il Senato non approva.**

che riguardano le banche dati. Ci sono alcuni sistemi, come CRIF e altri,

di queste banche dati private, che non sono della Banca d'Italia, è infinita. Per questa ragione chiedo l'attenzione del relatore, del Governo e dei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione,

del giorno G21.200, formulo un invito al ritiro perché venga tramutato nell'ordine del giorno con il contenuto dell'emendamento 21.202.

dell'ordine del giorno G21.200, perché ne condivido le motivazioni e non le ho sentite contestare

Mi spiace contraddire il collega Lannutti su questo punto, ma mi meraviglio che fino ad oggi banche dati private come Moody's, Standard & Poor's e Fitch siano state considerate cattedrali inoppugnabili.

di milioni di cittadini e di consumatori. Capisco che chi vuole assumere da monopolista il ruolo di rappresentante dei consumatori attraverso associazioni che non hanno mai dimostrato il vero peso quantitativo dei loro aderenti sia contrario all'uso di queste banche dati, ma personalmente credo che magari ce ne fossero altre - tutte quelle disponibili - per difendere il povero cittadino indifeso e la piccola impresa,

condizioni migliori e tassi d'interesse più

Do la parola al senatore Lannutti, ma è veramente difficile, colleghi, riuscire a seguire il dibattito

La materia è complessa ed è giusto quindi che il Governo, a fronte dei problemi che sono stati sollevati e che trovano tutta l'Assemblea concorde (non è dunque questione di maggioranza od opposizione),

senatore Lannutti),

Tale fenomeno corrode il tessuto sociale ed economico di vastissime aree del nostro Paese; in alcune realtà è un fenomeno storico e sedimentato, in altre è più recente ma ugualmente insidioso. Il *racket* delle estorsioni produce distorsioni gravi e drammatiche sia sul versante della sicurezza per i cittadini, sia su quello dello sviluppo economico. La sua carica distruttiva ha piegato e reso subalterni tanti operatori economici e intere generazioni di imprenditori. La povertà e la disoccupazione massicciamente presenti nel nostro Meridione hanno una loro origine nel ricatto estorsivo organizzato, fondamentale, a sua volta, per controllare capillarmente i territori da parte dei *clan* malavitosi e per foraggiare altre attività illecite. Tale fenomeno estorsivo è altresì divenuto strumento di controllo criminale del territorio e di penetrazione e di controllo del sistema economico anche fuori dalle Regioni meridionali. Nel settembre 2007 Confindustria Sicilia ha adottato un codice etico per i propri associati volto a scoraggiare e a punire ogni sorta di cedimento o di collusione con pratiche di carattere estorsivo. A seguito di un intensificarsi delle minacce e delle intimidazioni si è reso necessario, da parte degli industriali impegnati sempre più in circuiti competitivi internazionali, intervenire affinché un anello fondamentale dell'ingranaggio estorsivo venisse meno e così disinnescasse un sistema divenuto ormai cronico. Il libero mercato, la competitività, l'occupazione e l'iniziativa imprenditoriale sono elementi essenziali e propulsivi di una società organizzata. L'emendamento in questione, che sottoponiamo all'Assemblea, vuole accordare un vantaggio a quegli operatori economici che intendono collaborare con lo Stato denunciando i ricatti estorsivi di cui sono oggetto e che sono soggetti, a causa di tali ricatti, a conseguenze rese ancora più pesanti in ragione della dimensione modesta della loro attività. Rendere conveniente la denuncia, signora Presidente, è la risposta che la politica deve dare agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani che intendono sottrarsi al gioco della criminalità organizzata. Pertanto l'emendamento in titolo prevede particolari incentivi e agevolazioni economico-fiscali, che costituiscono un'implementazione dei sistemi di garanzia e di sicurezza per l'incolumità di chi denuncia e per la salvaguardia dell'attività economica di piccole e medie dimensioni e pertanto meno capaci di assorbire i contraccolpi

Non è la prima volta che accade ed è una sceneggiata continua.

per il quale bisogna dare atto al relatore, oltre che alla maggioranza ed al Governo, di un rapporto proficuo e di grande collaborazione con le opposizioni. Il testo che ci accingiamo ad approvare è stato sensibilmente migliorato grazie al lavoro svolto in Commissione ed in Aula. Esso tenta di dare una risposta, ancorché parziale, ad un problema che, a seguito della crisi economica e finanziaria globale e del nostro Paese... Mi scusi, senatore D'Alia. Colleghi senatori, come potete immaginare, il senatore D'Alia ha una certa difficoltà ad esprimersi in queste condizioni e ha una certa difficoltà anche la Presidenza a sentirlo. Prego, senatore Come dicevo, si tratta di una risposta, parziale perché ovviamente interviene solo su alcuni aspetti della materia, che si rende necessaria a seguito dell'aggravamento della situazione economica e finanziaria del nostro Paese, dovuto a ragioni sia che riguardano tutte il nostro Paese, sia che invece sono di natura più squisitamente congiunturale. cui viviamo, nel momento in cui lo Stato deve intervenire a sostegno delle banche per le note vicende, considerato che la situazione economica del Paese, come ammette anche oggi il nostro Presidente del Consiglio, è più grave e seria di quanto non sia stato apprezzato fino ad ora, tutto questo si scarica sul sistema economico delle famiglie e dei ceti deboli,

e che, quindi, in situazione di particolare crisi si trovano in condizioni di ulteriore svantaggio. Questo è l'*humus*, il terreno di coltura su cui si sviluppano i fenomeni legati all'usura. Questo è il terreno che aggrava anche la situazione nell'ambito della quale le organizzazioni criminali si muovono, ad esempio, con il reato di estorsione.

Parimenti è anche positiva l'altra parte dell'intervento che operiamo con il testo in esame, che riguarda l'introduzione di procedure che tendono a comporre, per le famiglie e per i singoli cittadini, i problemi legati al cosiddetto sovraindebitamento, che è un'altro terreno di coltura dell'usura.

criminali e la procedura che consente un minimo di sollievo alle famiglie che si indebitano, quando questo indebitamento, sopratutto in particolari momenti della vita economica del nostro Paese, è più alto.

importante, anche dal punto di vista simbolico, per rappresentare la immediatezza della pretesa punitiva dello Stato. Queste sono alcune delle considerazioni che ci permettiamo di svolgere. È chiaro che tutto ciò da solo non basta, perché non basta solo intervenire sulla legislazione penale e sulle procedure di concordato (perché, in senso lato, questo è anche la procedura che riguarda la composizione della crisi da indebitamento),

per il nostro sistema creditizio ed economico, ma oggi, nel momento in cui è ancora più difficile, per condizioni oggettive, l'accesso al credito, e le

che si sia intervenuti per effettuare alcune precisazioni, ma che sia altrettanto importante che noi ci si faccia carico di interventi legislativi che nel rapporto, che non è paritario, tra cittadino, impresa e sistema bancario, garantiscano di più il cittadino, l'impresa e le famiglie italiane, che sono i soggetti deboli, che vanno sempre e comunque maggiormente tutelati. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo parlamentare e ringrazio il relatore, i colleghi della maggioranza e il Governo che si sono fatti carico

lo è a scapito delle famiglie, delle piccole e medie imprese, di chi - l'ho già ricordato ieri - si deve impiccare perché non ce la fa a pagare, perché perde la casa,

nasce in banca, da un credito negato, dall'insensibilità del sistema bancario a valutare la meritorietà del credito. Signora Presidente, non voglio farla lunga. Pertanto, ringrazio ancora

questo archivio sono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario. Queste informazioni vengono rese disponibili per le banche al fine della valutazione dell'affidabilità

L'effetto di queste segnalazioni è quasi identico a quello delle segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia e spesso anche peggiori, perché per segnalazioni di lievissima entità l'utente si è visto poi negare finanziamenti ben più importanti, pur essendo pienamente solvibile. Di fronte a situazioni di erronee valutazioni delle condizioni dell'utente dei servizi bancari, che avevano dato luogo ad illegittime segnalazioni, vi sono state numerose pronunce giurisdizionali che hanno imposto alla banca, anche in via d'urgenza, di rettificare i dati che avevano dato luogo alla segnalazione, con cancellazione della segnalazione ed in alcuni casi con il risarcimento dei danni liquidati a favore del soggetto leso dal comportamento illegittimo.

impegnare il suo tempo in una sorta di *via crucis*. L'iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati, immotivata o conseguente ad erronee valutazioni o a segnalazioni di lievissima entità, in seguito alla quale colui che si rivolge ad una banca per avere un prestito si vede negare il credito, rappresenta l'anticamera dell'usura. Ricordiamocelo bene: l'anticamera dell'usura!

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, è perfettamente legittima la richiesta di coloro che, una volta sanata la morosità, pretendano la correzione dei dati della loro segnalazione non più attuale; tuttavia, nella maggior parte dei casi si verifica un'ostinazione da parte della banca dati alla non correzione di questi dati. Chiudo, signora Presidente, ribadendo il nostro

Non so se sia un caso, perché probabilmente il momento che stiamo vivendo crea le condizioni migliori perché il fenomeno continui, dilaghi, esploda.

imprese, di accesso al credito, oggi si aggiunge una grande crisi finanziaria, per cui o c'è una grande patrimonializzazione oppure il credito è spesso frenato o negato. il credito "legale", non resta che raggiungere il credito illegale o l'usura, che sono l'unica via di sfogo. Il fenomeno è conosciuto. Queste Aule hanno hanno affrontato l'argomento in più legislature, con Commissioni parlamentari che hanno sviscerato il problema e lavorato in modo serio.

la dimensione reale di questo problema. È chiaro che si doveva stabilire che chi era soggetto ad usura doveva essere vittima stimolata a denunciare, pertanto tutelata successivamente dal nostro ordinamento. A dieci anni dall'ultima riforma in materia, era sicuramente necessaria una manutenzione del sistema. Come Lega volevamo però porre l'attenzione sulla seconda parte di questo provvedimento, una procedura molto snella che, con l'avallo dei creditori, istituisce una sorta di concordato per debiti per lo più contratti per necessità o da microimprese o da autonomi

A noi piace perché intervengono organi tutori e di garanzia. Gli organismi per la compensazione della crisi sono di due specie, ambedue istituzionali, tanto gli organismi di conciliazione presso le Camere di commercio quanto gli ordini

verificare quanto è possibile recuperare. A volte i crediti sono difficilmente esigibili al momento, però il creditore potrebbe attendere quel tanto che basta per veder soddisfatti i propri diritti piuttosto che perdere sostanzialmente tutto.

È interessante capire quali garanzie esistono; infatti, è depositato presso il tribunale tutto l'elenco dei creditori, con tutte le somme a credito e tutte gli atti dispositivi e retroattivi di cinque anni. D'altra parte,

opera non con il classico sistema della notifica e del formalismo, ma con ogni forma di comunicazione: può inviare lettere, telegrammi o telefax; l'importante è che vi sia un sistema che arrivi a comunicare.

Oggi parliamo della tutela di un'ipotetica vittima dei clan dell'usura, però non possiamo perdere di vista i sacrosanti diritti di un creditore, che potrebbe essere esposto a rischio

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il disegno di legge in materia di lotta all'usura e all'estorsione merita una particolare attenzione, trattandosi di illeciti odiosi e destabilizzanti per la serenità dei nostri concittadini che si trovano in condizioni di sovraindebitamento. L'aggiornamento normativo proposto promana senza dubbio alcuno da una ineludibile esigenze evolutiva, anche per i tempi di crisi economica che viviamo. Certamente il provvedimento andrà ad incidere positivamente, in termini di sostegno, su quelle famiglie che per vicende varie si trovano in una situazione di grave disagio economico. Il contesto più impegnativo su cui si vuole e si deve intervenire è però quello criminale, in particolare nei territori a più elevato tasso di mafiosità, ed è dunque auspicabile che le necessarie riflessioni sull'argomento possano condurre a sollecitazioni rivolte a tutto il settore del credito legale, che proprio in quei territori dovrebbe assumere un autorevole e chiaro atteggiamento collaborativo e di sostegno, abbandonando prassi quantomeno arroganti, recentemente richiamate anche dal Governatore della Banca d'Italia, spingono inesorabilmente a rivolgersi al mondo dell'usura. Su questo punto il senatore Lannutti è stato quanto mai esplicito. Devo osservare che da tempo seguo un contenzioso giudiziario tra un imprenditore calabrese ed alcuni istituti di credito. La sentenza di primo grado ha confermato che l'imprenditore è stato vittima di usura, ma non sono stati individuati gli autori ed è significativo che nella prima udienza in corte d'appello è stata disposta la riapertura dell'istruttoria: sarà interessante conoscere le conclusioni del processo. Proprio sulla base di queste considerazioni il provvedimento all'esame dell'Assemblea ha anche un'altra importante caratteristica, oltre a quella di una migliore incisività sul fronte del contrasto alla criminalità mafiosa: infatti sul fronte della prevenzione in generale, sollecitando controlli più puntuali e migliori *performance* della pubblica amministrazione, specialmente in termini di flessibilità e di semplificazione. Dagli interventi in discussione generale, del relatore senatore Mazzatorta, del senatore Lauro, del senatore Lumia e della senatrice Della Monica, emerge una chiara condivisione dell'impianto della norma, a significare che non ci sono dubbi: il fronte è comune e la strategia può essere concertata e quindi condivisa. È un auspicio che mi appartiene e che ha sempre caratterizzato la mia attività istituzionale nei vari incarichi che ho avuto il privilegio di svolgere.

Le modifiche delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 intervengono non solo in modo sostanziale sulle procedure, sui requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche sul ruolo delle associazioni, che saranno più puntualmente selezionate con il decreto del Ministro dell'interno. Significativo è anche il recupero dell'imprenditore fallito e altrettanto interessanti sono le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,

Condivisibile è l'innovativo procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, con l'individuazione di organismi di composizione che dovranno esercitare il ruolo con una chiara assunzione di responsabilità. Inoltre, è interessante rilevare come questo provvedimento si inserisca in uno degli obiettivi prioritari programmati dall'attuale Commissione parlamentare antimafia in sede propositiva: la collocazione sistemica delle normative antimafia in un Testo unico, in modo da consentirne anche un'agile applicazione. Certamente, la normativa in materia di lotta all'usura e all'estorsione, così aggiornata anche se migliorabile, potrà far parte del contesto unitario insieme ad altre rilevanti norme, quali quelle relative alla certificazione antimafia, ai beni sequestrati e confiscati, allo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa, al trattamento dei rifiuti, al testimone di giustizia, ovviamente tenendo presente che l'elenco non è esaustivo. Queste norme meritano, comunque, una particolare attenzione in termini di aggiornamento Tutto ciò conduce inesorabilmente al concetto di sicurezza sistemica, che è la sfida vera vera che la politica e la pubblica amministrazione, nonché questo Parlamento, devono raccogliere e saper vincere, tenendo presente che sicurezza sistemica significa assunzione di responsabilità e rispetto delle competenze e dei ruoli; significa esercitare autorevolezza e non autoritarismo; significa che forze di polizia e magistratura hanno sì responsabilità esclusive nell'esercizio delle specifiche funzioni sul fronte del contrasto della criminalità organizzata, ma sono concorrenziali su quella della prevenzione generale, laddove si esigono le migliori *performance*, specialmente da parte del mondo politico. La mia esperienza istituzionale mi ha consentito, nel mio penultimo incarico a Reggio Calabria, di assumere tutte le responsabilità che mi competevano e di cercare di dare le risposte più esaustive possibile alla cittadinanza. Una sola volta mi sono trovato in imbarazzo istituzionale, quando un imprenditore che aveva reiteratamente denunziato i vari tentativi di estorsione venne a rappresentarmi il suo vivere e quello della sua famiglia e mi pose una sola domanda: la libertà di lavorare. Ritengo che oggi, varando il disegno di legge in esame, abbiamo abbattuto di quale punto percentuale questo imbarazzo istituzionale. Per questi motivi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento. *(Applausi

MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che oggi in quest'Aula si stia dando la più convincente dimostrazione dell'essenzialità del ruolo e delle funzioni parlamentari e parimenti, al di là di ogni strumentale polemica, della forte interazione che sussiste e intercorre tra Parlamento e Governo. Trattasi infatti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare dei colleghi Centaro e De Lillo (i due disegni di legge sono stati accorpati), che grazie al proficuo lavoro della Commissione di merito e di quest'Aula

introducendo previsioni che più adeguatamente, nel relativo meccanismo sanzionatorio, diano contezza dell'elevatissimo disvalore sociale delle condotte sanzionate, adottando strumenti processuali che più adeguatamente garantiscano che, nel rispetto dell'inalienabile diritto alla difesa, siffatto sistema sanzionatorio possa trovare concreta applicazione. Parimenti, onorevoli colleghi, in linea con gli altri grandi ordinamenti europei abbiamo affrontato con grande senso di responsabilità e realismo le drammatiche conseguenze che sul piano economico e sociale siffatte condizioni delittuose determinano; non solo migliorando la normativa già in vigore, che prevede interventi ed agevolazioni in favore di quanti, vittime di tali odiosi reati, versano in gravissime condizioni economiche, altresì introducendo, attraverso il prezioso lavoro prima della Commissione e poi dell'Aula, innovativi strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento che, sia pur nel solco di una rigorosa tutela delle ragioni dei terzi onesti creditori, consenta a tali vittime finalmente di uscire dal lungo incubo nel quale sono vissute, dando loro la speranza e la possibilità di una vita normale. Concludendo, colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, mi sento di affermare che oggi questo ramo del Parlamento, assolvendo e ribadendo la sua essenziale funzione, ha scritto una pagina virtuosa della storia parlamentare, aggiungendo un prezioso tassello a quel percorso di recupero del rapporto tra cittadini e istituzioni che è il fondamentale collante di ogni grande Nazione civile.

il Senato approva

già prevista dal calendario per la seduta antimeridiana di domani, è anticipata alla seduta pomeridiana di oggi, che pertanto potrà perseguire anche oltre le ore 20.

sul Governo afgano affinché sia abrogata la legge approvata qualche giorno fa da quel Parlamento, che permette lo stupro delle donne da parte dei mariti o degli amici in casa e che non permette alle donne afgane di uscire di casa per andare dal medico senza il il permesso del marito. Che l'Europa prenda posizione, ricordando che solo l'Italia negli ultimi due anni ha versato 600 milioni di euro, 13 soldati morti e che stiamo inviando altri 250 militari italiani per intervenire in difesa delle elezioni libere in quel Paese. Ritengo che abbiamo tutti gli strumenti, signora Presidente, per intervenire in difesa delle donne.

la situazione venutasi a determinare nelle carceri per la mancanza di psicologi. Purtroppo questa notte la mancanza di psicologi ha fatto un'altra vittima:

sta diventando drammatica. I livelli di assistenza che l'amministrazione penitenziaria è in grado di assicurare, infatti, sono di gran lunga al di sotto di quelli che possono essere considerati civili, come peraltro lo stesso Ministro in più occasioni ha sostenuto. Purtroppo è in aumento il tasso di suicidi e, addirittura, l'ultimo caso verificatosi ieri assume un ulteriore connotato di gravità, perché la persona in questione, in assenza di psicologi nel carcere di Marsala era stata vista da un medico, e poco dopo, rientrata in cella, si è impiccata. Tutto ciò costituisce un ulteriore elemento aggravante di una condizione che non può più essere trascurata. Il sovraffollamento, l'inadeguatezza delle strutture, l'assenza di personale specializzato, con particolare riferimento agli psicologi, le difficoltà con cui la sanità penitenziaria si sta trasferendo al Servizio sanitario nazionale, costituiscono un quadro essenziale del dramma delle nostre carceri, che stanno diventando - e concludo, Presidente, scusandomi per essermi dilungato - delle bombe ad orologeria.